Vedo il senatore Di Lello presente in Aula, mi associo agli auguri, ma vedo che non ne ha troppo bisogno. *(Applausi

per comodità di tutti riepilogo quello che sarà l'andamento dei nostri lavori nella giornata odierna. In primo luogo, come convenuto, passeremo all'esame del decreto-legge recante disposizioni in materia tributaria e finanziaria. per primi i relatori Legnini e Benvenuto; si passerà poi all'illustrazione delle questioni pregiudiziali (una delle quali è già stata presentata) e delle eventuali sospensive. Si svolgerà quindi un'unica discussione su tutte le proposte, nel corso della quale potrà intervenire, Sempre in base al Regolamento, sarà quindi effettuata una votazione per le diverse questioni pregiudiziali, ed una per le eventuali sospensive. Conclusa questa fase, si riprenderà con l'esame degli articoli e degli emendamenti della Legge comunitaria.

al fine di individuare un meccanismo diverso per affrontare la discussione della legge finanziaria. C'è un continuismo negli ultimi quattro anni che porta a una discussione convulsa, a una discussione nella quale il ruolo del Parlamento è oscurato dal sovrapporsi e dal rincorrersi delle posizioni. Da qui la necessità di una riflessione che ci permetta, d'ora in avanti, di affrontare la legge finanziaria in una logica nella quale sia esaltato e valorizzato il ruolo del Parlamento. In secondo luogo, il decreto-legge che dobbiamo convertire e che ci è venuto dalla Camera rientra nella manovra di politica economica, che secondo la maggioranza e secondo l'Unione, ha come punti di riferimento lo sviluppo, il rigore e l'equità. Siamo convinti che occorra operare il rientro nei parametri di Maastricht secondo gli impegni che erano stati presi dal precedente Governo e siamo convinti che tale operazione, che indubbiamente ha un peso rilevante, comporti problemi nella definizione della manovra di politica economica, perché deve riuscire a realizzare un collegamento tra lo sviluppo e il rigore - ma non una politica indiscriminata di tagli - e creare le condizioni perché tale operazione non ignori i problemi dell'equità. esponenti dell'opposizione: ma questa operazione poteva essere fatta in più di un anno. No, è importante che l'operazione venga fatta

ci devono far riflettere i segnali che vengono dalle società di *rating*. Essa deve permetterci di cogliere l'opportunità di una ripresa che si sta manifestando in Europa e che vede anche l'Italia interessata; farla in un anno

la stagione delle riforme strutturali di cui ha bisogno il nostro Paese per tornare ad essere competitivo; libererà l'Italia dall'angoscia che ha conosciuto il Governo di centro‑destra quando, nella passata legislatura,

manifestata una linea dell'opposizione radicalmente diversa da quella della maggioranza: una linea che ha puntato esclusivamente ad un'operazione di tagli,

di tagli della spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge per spese obbligatorie ed interessi sui titoli del debito pubblico. Una linea, questa, radicale, radicale, che toglieva il giusto, ma che toglieva anche ciò che non è giusto; una linea che, a nostro avviso, non si sostanziava e non garantiva al Paese né l'equità né lo sviluppo. Ancora, l'opposizione ha posto altri problemi alla base dei suoi emendamenti e della sua scelta strategica,

tagli alla cooperazione e al fondo spettacolo e cultura, tagli al trasporto pubblico, tagli alla messa in sicurezza delle nostre sedi all'estero o addirittura il taglio del 90 per cento dei trasferimenti correnti alle imprese. Noi non abbiamo condiviso questa linea e abbiamo invece difeso la sostanza e il cuore del nostro provvedimento, del decreto‑legge, che ha al centro, come elemento fondamentale, la lotta e l'azione di contrasto all'evasione fiscale. Abbiamo puntualizzato, in primo luogo, che la lotta all'evasione fiscale è un interesse e una necessità per il nostro Paese.

per diminuire la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Come si realizza tale operazione? Anche a

e della Guardia di finanza per svolgere operazioni di contrasto al problema della contraffazione e a quello delle merci che invadono il nostro Paese. Si tratta di misure specifiche

Tutti sappiamo che tale sistema è stato per anni il tallone d'Achille del nostro sistema fiscale: si accertava 100, si incassava 5, costava 6.

le misure, che erano già state previste in quello scorcio della passata legislatura, vengono rafforzate e definite. Già quest'anno possiamo raccogliere

nella lotta all'evasione fiscale è data dalla realizzazione del passaggio e del lavoro comune a proposito del catasto. Anche qui, nella passata legislatura, si era andati di proroga in proroga, anche se nell'ultima legge finanziaria erano stati fatti passi in avanti, responsabilizzando e facendo...

sta dando dei risultati e permetterà, con le decisioni pratiche che sono contenute nel decreto, di introdurre degli elementi di equità e di razionalizzazione

Con quest'opera di razionalizzazione, che vede già il pagamento dell'ICI su edifici che hanno perso le loro caratteristiche originarie (penso agli immobili cartolarizzati, a quelli delle grandi stazioni, dei grandi aeroporti e dei porti, agli edifici che hanno perso le caratteristiche di ruralità), si trovano le risorse per compiere un'operazione di carattere equitativo tale da permettere di intervenire sull'ICI come prima abitazione per i redditi più bassi.

tra costi e ricavi e nei costi si possono detrarre una serie di spese. È proprio per venire incontro al fatto che il reddito da lavoro dipendente verrebbe tassato, come del resto da noi, solo sui ricavi, che negli Stati Uniti

positivo nelle ristrutturazioni abitative. Si possono compiere limitati approfondimenti, si può esplorare, ma la vera lotta all'evasione fiscale rientra in quelle scelte e anche nelle decisioni che già sono state prese

che tale condono valeva a partire dal pagamento della prima rata, si sono dimenticati di pagare le rate successive. In secondo luogo, si è intensificato il controllo su quelle aziende che non hanno occupati, che non producono se non fatture false. Si è quindi intervenuti sulla cosiddetta IVA carosello e, ancora, sono state previste delle norme più stringenti per quanto riguarda il problema delle compensazioni. Questo Questo è il cuore della politica fiscale. Ci sono poi delle questioni affrontate nel decreto-legge che non abbiamo avuto la possibilità di modificare. Noi, come maggioranza, sin dall'inizio del dibattito abbiamo precisato che non sarebbero stati presentati emendamenti e abbiamo concentrato la nostra azione nella predisposizione di alcuni ordini del giorno

Prego, senatore Benvenuto.

riservare una considerazione particolare per gli eredi portatori di *handicap*; abbiamo poi posto il problema di chiarire bene il regime che si individua per il terzo settore e per le ONLUS;

Abbiamo presentato anche altri ordini del giorno per chiedere un impegno preciso da parte del Governo per quanto riguarda il regime della detrazione IVA che dovrà essere modificato alla luce delle intese che saranno raggiunte con l'Unione Europea dopo la nota sentenza di condanna del nostro Paese.

anche una scelta coraggiosa, quella di rifondare il rapporto tra amministrazione, istituzioni e cittadini su un piano di fiducia e collaborazione.

sarebbe infantile. Ecco perché rappresentiamo al Governo, con un ordine del giorno preciso, la necessità che lo Statuto dei diritti

Pensiamo infatti che la necessaria lotta all'evasione fiscale richieda una grande capacità preventiva, ancor prima che repressiva, che possa consentire, con la collaborazione di tutti, di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale. Infatti, l'evasione fiscale non è solo un fenomeno di profonda iniquità, è anche un problema grave di mortificazione della professionalità e di alterazione della concorrenza nel mercato. Ecco perché gli ordini del giorno vanno in quella direzione, ecco perché riconfermiamo il grande valore della scelta della lotta all'evasione fiscale. Ecco perché, in conclusione, diciamo ai colleghi dell'opposizione che parlano di «grande fratello» che qui non c'è un grande fratello, c'è una grande evasione che richiede l'impegno, la collaborazione e lo sforzo di tutti per essere debellata e sconfitta.

Spesso si sono confrontati due punti di vista in modo chiaro e lineare, alternativi sulla politica economica e finanziaria, sulla politica fiscale

le misure proposte e ad enfatizzarne l'efficacia e gli effetti in modo negativo, degradando, in alcuni casi, in allarmismi inutili ed ingiustificati.

senza sottrarci al confronto sui temi di carattere più generale, di ricondurre comunque al merito del provvedimento la discussione che abbiamo tenuto, tenuto, rivendicando la coerenza del decreto stesso con l'impostazione complessiva di politica economica e di bilancio tracciata tracciata nel Documento di programmazione economico-finanziaria nel luglio scorso, un documento che aveva l'ambizione di essere, appunto, di legislatura. Abbiamo altresì affermato ed affermiamo che il risanamento dei conti pubblici è una necessità per il nostro Paese e lo è non solo perché ce lo impone l'Europa, ma perché l'eredità e gli gli effetti delle politiche di questi anni sono molto pesanti. Come è noto a tutti, il debito è tornato a crescere negli ultimi due anni, collocandosi al 107,7

L'avanzo primario è stato praticamente azzerato: dal 5,5 per cento del PIL nel 2000, si è ridotto allo 0,4 per cento del PIL nel 2005; l'indebitamento delle pubbliche amministrazioni è cresciuto del 3,3 per cento nel quinquennio; il rapporto *deficit*-PIL si è attestato quest'anno al 4,1 per cento, collocandosi ben oltre i parametri imposti dall'Unione Europea e ben oltre le previsioni contenute nella manovra finanziaria dello scorso anno. Gli effetti della nota sentenza sulla detraibilità dell'IVA sulle autovetture ha ulteriormente aggravato il quadro di finanza pubblica. La manovra di correzione non poteva, quindi, limitarsi ad un mero aggiustamento, come invocato dai nostri oppositori: occorreva ed occorre invertire la tendenza sul fronte dei conti pubblici; ricondurre i saldi entro i limiti che ci sono imposti e che ci siamo prefissati con il DPEF; ricominciare a ricostruire l'avanzo primario, che costituisce la vera fonte di virtuosità della politica di bilancio e far tornare a scendere il debito. Sono questi gli obiettivi principali della manovra, relativamente all'obiettivo del risanamento dei conti, ai quali si aggiunge, come è noto a tutti, la necessità di reperire risorse per soddisfare le politiche di equità I margini per conseguire l'obiettivo del risanamento erano e sono ristretti, come abbiamo sottolineato più volte. Il ventaglio delle opzioni a nostra disposizione, in virtù dei vincoli e delle rigidità del bilancio pubblico, ulteriormente aggravati in questi anni, è alquanto ridotto. Puntare, come ci è stato detto, tutto sulla riduzione di spesa era ed è irrealistico, almeno nel breve periodo il fallimento delle politiche di questi anni ne costituisce la dimostrazione: riduzioni di spesa invocate e normate sono state, molte volte, soltanto virtuali. Occorreva, quindi, puntare sui risparmi, ma in modo realistico. E i risparmi in questa manovra finanziaria ci sono. Ci sono riduzioni ragionate e concertate sul sistema degli enti locali, sui Ministeri; vi è uno sforzo di riduzione di sprechi, di enti e vi è un taglio della spesa tendenziale sulla sanità, seppur nel contesto di una crescita nominale della spesa sanitaria. Ma per conseguire obiettivi più ambiziosi - lo abbiamo detto - occorrevano ed occorrono riforme incisive e strutturali, in particolare sul sistema pensionistico, sul pubblico impiego, sull'assetto e l'efficienza delle amministrazioni centrali. Obiettivi che intendiamo conseguire nel prossimo futuro e che daranno frutti, in termini di risparmio di spesa, nel medio-lungo periodo. La nostra sfida, la sfida di questa maggioranza, nel prossimo futuro, è esattamente questa, sulla linea tracciata

precedenti il vostro Governo. Voi, che vi siete dichiarati alfieri dei tagli di spesa, avete realizzato il cosiddetto

L'altro pilastro del risanamento è - come ha ampiamente annunciato il presidente Benvenuto - un regime di tassazione più equo e ripulito dai mali dell'evasione e dell'elusione fiscale. Questo è l'obiettivo principale del provvedimento al nostro esame: apprestare una parte importante delle risorse per sostenere la manovra finanziaria, per contribuire ai risultati della stessa, per invertire la tendenza sul fronte dell'evasione e dell'elusione, per completare la strumentazione a tal fine necessaria, che era già stata

- sull'esigenza, che poniamo, di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, ma nulla hanno proposto di alternativo rispetto alle misure contenute nel decreto-legge,

una politica di riduzione della pressione fiscale, ottenendo però un risultato impercettibile (qualche decimale di punto di riduzione della pressione fiscale), ma nel contempo stressato il bilancio dello Stato, deprimendo il sistema economico. Quest'anno, nel 2006, è bene ricordarlo, con la con la vostra finanziaria, la pressione fiscale è destinata ad aumentare dello 0,8 per cento; nel 2007, con questa manovra finanziaria, ci sarà sì un incremento della pressione fiscale, ma ben inferiore a quello del 2006, dello 0,4-0,5 per cento, al netto delle entrate relative alla misura sul TFR, che non si può dire finalizzata ad aumentare la pressione fiscale stante la natura della misura medesima. Questi sono i dati e non quelli che vengono urlati in questi giorni. Il confronto si è compendiato su questo punto, alla fine della discussione, su due obiettivi che riteniamo immediati,

approvato questa notte in Commissione, la inderogabilità e l'esigenza del rispetto dello Statuto del contribuente, che è stato troppe volte violato anche nella passata legislatura. Vogliamo che le risorse aggiuntive provenienti dal contrasto all'evasione fiscale siano finalizzate alla riduzione della pressione fiscale, come già indicato nella risoluzione conclusiva sul DPEF, e lo vogliamo fare con una innovazione importante, incidendo direttamente, possibilmente, sull'articolo 1 della finanziaria, in modo tale da prefigurare un meccanismo automatico che è difficile, ma possibile normare. In tal modo, riteniamo di poter conseguire quegli obiettivi di equità e di contributo al risanamento cui mi riferivo prima. Il confronto nelle Commissioni è stato comunque improntato alla chiarezza. Noi abbiamo posto due esigenze: una, quella di approvare sollecitamente questo decreto, che ha un rapporto stretto con la manovra finanziaria per le ragioni a cui accennavo prima; un'altra, quella di raccogliere gli elementi più importanti provenienti dalla discussione e di impegnarsi ad apportare correzioni e integrazioni con la discussione che effettueremo nelle prossime settimane sulla legge finanziaria. L'opposizione, nella fase conclusiva della discussione, si è sottratta La maggioranza, invece, ha approfondito in modo serio i temi posti dal dibattito, conseguendo risultati importanti affidati alla stesura e all'approvazione di diversi ordini del giorno, che hanno un contenuto preciso e impegnativo, e che potranno contribuire a migliorare le misure che oggi stiamo discutendo. Si tratta di ordini del giorno non formali, non approvati tanto per approvarli, ma per dare indicazioni concrete alla maggioranza e all'intero Parlamento sulle direttrici di miglioramento che vogliamo conseguire con la discussione sulla legge finanziaria. Lo abbiamo fatto per la parte fiscale e anche per la seconda parte del decreto, che affronta problemi urgenti e importanti: le problematiche della finalizzazione delle risorse già assegnate alla prima fase di realizzazione dello Stretto di Messina, oggetto di discussione e, appunto, di una indicazione precisa, seppur generale, in un ordine del giorno; lo abbiamo fatto sul riordino importante degli enti di ricerca, prevedendo nel decreto l'istituzione di un nuovo unico ente che dovrà sovrintendere alla valutazione della ricerca sostituendo i diversi enti esistenti; lo abbiamo fatto sul tema dell'editoria, prevedendo il riordino della disciplina; lo abbiamo fatto sullo *spoils system* e su altre norme. Ma lo abbiamo fatto soprattutto su un tema centrale e importante di questo decreto, quello che riguarda l'ANAS e le concessioni autostradali. Gli obiettivi delle norme contenute nel decreto erano e sono chiari: rendere più efficaci e rispondenti all'interesse pubblico le numerose convenzioni in essere (che sono state stipulate nel corso degli anni e si sono sovrapposte, anche attraverso numerose revisioni stipulate, appunto, negli anni); cogliere le revisioni periodiche previste nelle convenzioni in essere per pervenire alla stipula di una convenzione unica (il decreto indica gli obiettivi della convenzione unica, ma la stessa dev'essere ancora redatta, poi dovrà passare al vaglio del CIPE e delle Commissioni parlamentari); rafforzare gli obblighi sugli investimenti; rendere effettive le sanzioni che sono già previste; ristabilire un rapporto serio tra il sistema tariffario,

dalle società concessionarie; introdurre, recependo in tal modo precise direttive europee, princìpi di concorrenza, attraverso l'eliminazione di quel di quel limite alla partecipazione alla società concessionaria autostradale imposto alle società di costruzione e rendendo altresì obbligatorie le gare pubbliche per gli appalti di lavoro e di servizi Il punto critico che abbiamo affrontato - mi avvio a concludere - riguarda l'incidenza delle nuove norme sui contratti in essere, che, com'è noto, hanno natura privatistica; su questo punto si sono contrapposte due posizioni, non solo nella discussione, ma anche nel Paese. Una posizione ritiene che l'interesse pubblico, che le norme di cui stiamo discutendo intende soddisfare, sia tale da poter incidere sulla rinegoziazione dei contratti in essere, prevedendone non soltanto il carattere ricognitivo, ma anche la modificazione in rapporto alle nuove regole. L'altra posizione asserisce una violazione dei princìpi costituzionali e dei princìpi di libera concorrenza e libera circolazione dei capitali; su questo punto, l'altro ieri, è stata avviata una procedura da parte della Commissione europea. Noi non ci siamo sottratti all'esigenza di affrontare questa problematica; abbiamo discusso e abbiamo predisposto un ordine del giorno chiaro, che ci consente di avviare, nel prossimo discussione finalizzata eventualmente a riesaminare talune norme sul punto specifico a cui mi riferivo prima (in rapporto all'esito della procedura avviata dalla Commissione Mi scusi, senatore Legnini. imponiamo ai relatori la necessità di una capacità di concentrazione fuori dal comune; non so come facciano. Chiedo quindi rispetto per gli altri. Vada avanti, senatore nel periodo di attuazione della nuova normativa. Su molti altri temi abbiamo formulato proposte e approvato ordini del giorno. Il prosieguo del confronto ci consentirà, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, di tradurre quelle indicazioni in norme da inserire nella finanziaria o in altri provvedimenti successivi. Signor Presidente, ho già detto all'inizio che intendiamo approvare questo decreto, approvarlo rapidamente, perché esso fornisce risorse, fornisce certezza al contenuto della manovra finanziaria nel suo complesso, ne anticipa alcuni contenuti, sostanzia, come mai è avvenuto prima, un equilibrio tra risparmi di spesa, quelli possibili, quelli realisticamente conseguibili, e nuove entrate, ci consente di guardare al futuro non solo della finanza pubblica, ma del Paese, della nostra economia con maggiore fiducia e con serenità.

Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, in data 29 settembre 2006, il Governo ha emanato il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ora in discussione per la conversione in questo ramo del Parlamento. I commi 159, 160, 161 e 162, già contenuti in qualche parte delle disposizioni all'articolo 41 del decreto-legge, che oggi fanno parte dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge e che riguardano la disciplina degli incarichi dirigenziali sono, a nostro giudizio, in palese contrasto con la Costituzione. Innanzitutto, le disposizioni del comma 161,

In particolare, il comma 161 introduce un meccanismo di *spoils* *system* totalmente automatico, che è ben più gravoso di quello previsto dalle precedenti disposizioni (che pure hanno dato luogo a diverse ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in attesa di essere decise), in quanto prescinde da qualsiasi valutazione dell'operato del dirigente e, oltretutto, estende in modo considerevole il suo campo di applicazione. A quest'ultimo riguardo va ricordato che l'articolo 19, comma 8, nella sua originaria formulazione, prevedeva l'applicazione dello *spoils* *system* ai soli soggetti che rivestano posizioni apicali, ossia il segretario generale dei Ministeri e il capo dei dipartimenti, mentre l'attuale comma 161 lo estende anche nei confronti di dirigenti di livello non apicale. In tal modo, da un lato vengono accomunate posizioni soggettive profondamente diverse,

che vieta di trattare nello stesso modo situazioni non assimilabili; dall'altro, nei confronti dei nuovi soggetti ai quali viene esteso lo *spoils* *system*, quest'ultimo risulta ancora più ingiustificato in quanto essi non occupano nemmeno incarichi apicali per i quali sia, al limite, ipotizzabile la necessità di uno stretto vincolo fiduciario con il Governo. I commi 159, 160 e 161 e 162 violano, altresì, l'articolo 97 della Costituzione in quanto essi prescindono da qualsiasi valutazione delle concrete ed effettive esigenze delle singole strutture amministrative nelle quali quei dirigenti sono o saranno inseriti, e più in generale prescinde da qualsiasi valutazione dell'impatto specifico che la rimozione di ciascun dirigente può provocare sull'andamento efficiente dell'amministrazione stessa. Inoltre, le predette disposizioni violano il principio del buon andamento, oltre che per la ragione ora evidenziata, anche perché inficiano irrimediabilmente ogni garanzia di autonomia dei dirigenti, che è invece presupposto indispensabile perché ad essi sia consentito un esercizio imparziale delle loro funzioni, a sua volta necessario per assicurare l' imparzialità della pubblica amministrazione. Il comma 161, inoltre, è illegittimo perché contrasta anche con tutti i princìpi cosiddetti lavoristici della nostra Carta costituzionale (articoli 3, 4 e 35), che assicurano la stabilità dei contratti individuali di lavoro e, in ogni caso, vietano l'interruzione ingiustificata dei contratti stessi. Il comma 161, infatti, prevede una cessazione dall'incarico *ope* *legis*, senza alcuna giustificazione concreta né di tipo oggettivo, né di tipo soggettivo. La norma non fa alcun riferimento né alle esigenze delle strutture amministrative in cui i dirigenti sono inseriti, né alle loro attitudini e capacità professionali, né, tantomeno, alla verifica del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati. Il comma 160, che dispone la cessazione degli incarichi dirigenziali anche per i direttori delle Agenzie, incluse quelle «fiscali», istituite con decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha loro riconosciuto la più ampia autonomia operativa, avendo un proprio bilancio e operando sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni, è illegittimo perché non è coordinato con la disposizione prevista dall'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, che disciplina in modo differente la stessa materia. Un richiamo in tal senso è contenuto specificatamente nel *dossier* predisposto dall'Ufficio studi del Senato, rimasto finora inascoltato. Il comma 159 del decreto‑legge in esame non appare chiaro, considerato che l'inciso in esso contenuto «limitatamente al personale non appartenente a ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001», dà luogo a differenti e divergenti interpretazioni. Anche tale aspetto viene segnalato ugualmente inascoltato, nel predetto *dossier*. Infine, le disposizioni di cui sopra configurano un eccesso di potere legislativo e, di conseguenza, violano l'articolo 70 della Costituzione. Infatti, se il Parlamento convertisse il decreto-legge in legge, quest'ultima avrebbe gli effetti propri di un atto amministrativo o negoziale (revoca dell'incarico e/o licenziamento), in contrasto anche con il principio della distinzione del potere legislativo dal potere amministrativo.

In sostanza, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, e in conclusione, con la nuova disciplina dei commi 159, 160, 161 e gravemente colpito il principio di separazione tra politica e amministrazione, che è alla base dell'intera riforma di privatizzazione del pubblico impiego e che è stato ribadito dal decreto legislativo n. 165 del 2001, determinando una inevitabile politicizzazione della dirigenza. Ricordo ciò soprattutto al presidente Ciampi. Quando egli

ribadiamo quanto detto nelle competenti Commissioni, cioè che non vogliamo fare ostracismo rispetto a questo provvedimento, importante perché collegato alla legge finanziaria. Abbiamo però il dovere di correggere gli errori costituzionale, che sono evidenti e sui quali richiamiamo l'attenzione di tutti i colleghi, ovviamente, ma soprattutto degli ex Presidenti della Repubblica, che sono stati e devono essere, anche in questo difficile momento della vita del Paese, tutori della legittimità costituzionale delle leggi. Concludo con un ricordo, presidente Ciampi. Noi approvammo nella passata legislatura la legge sull'ordinamento giudiziario dopo una battaglia terribile. Quando lei dovette dare il parere sulla legittimità del provvedimento, lo rinviò,

per sé. Concludo ricordando che, quando si tratta di «legittimità illegittimate» di una norma, non vi è più distinzione fra maggioranza ed opposizione, ma vi è il dovere del Parlamento di evitare illegittimità.

le mie osservazioni, che riguardano pur sempre questioni di legittimità costituzionale, si traducono in una richiesta di sospensiva di due settimane

Alcune riguardano i presupposti, di cui abbiamo discusso; altre, invece, la sostanza del provvedimento. Il collega Saporito ne ha indicata una estremamente importante e delicata.

che cercano di intervenire sulle concessioni già definite e già storicamente consolidate appunto con norme di legge, contravvenendo a qualsiasi a qualsiasi rispetto dei patti che anche il legislatore e lo Stato devono, comunque, osservare. Si tratta di un aspetto molto delicato: se ne riparlerà nel merito, ma bisogna fin d'ora cogliere il lato di profonda illegittimità costituzionale che riguarda tali normative. Il secondo punto, Presidente, non meno importante, concerne la reintroduzione dell'imposta di successione. Voglio ricordare ai colleghi che dapprima il Governo tentò, il decreto-legge, di reintrodurla in maniera surrettizia, ipocrita diciamo, aumentando le imposte ipotecarie e catastali, introducendo un'imposta di registro. Alla fine, visto che il giochino di occultamento non riusciva, ha gettato la maschera e ha reintrodotto l'imposta di successione. Perché parlo di incostituzionalità? Perché nello Statuto del contribuente - mi riferisco al presidente Benvenuto che lo ha citato - vi è una disposizione precisa, precisa, che vieta di introdurre nuove imposte con decreti-legge. Questa norma certamente può essere superata dal legislatore ordinario con una norma in deroga,

comunque si lasciava un minimo di esenzione per i piccoli patrimoni e per le liberalità fatte anche in favore di estranei, di soggetti non legati da vincoli di parentela, magari di soggetti legati da vincoli affettivi o di riconoscenza. Vi era questo meccanismo

che richiede una riflessione - e mi fa piacere che ci sia la senatrice a vita Levi-Montalcini - riguarda la ricerca. Credo quindi che sarebbe opportuno un minimo di attenzione.

Proprio oggi, su uno dei rari giornali che sono in edicola, vi è un comunicato che riguarda il Consiglio universitario nazionale, il CUN. In questo comunicato, il CUN solleva fondati dubbi di legittimità costituzionale dei commi da 138 a 145 dell'articolo 2 di questo decreto-legge, perché ritiene che il rinvio a regolamenti di delegificazione violi una riserva di legge prevista dell'articolo 33 della Costituzione. Si dice infatti: «Gli enti di ricerca verrebbero controllati non più da leggi ma da semplici regolamenti, con i quali potrebbero anche essere soppressi, fusi, istituiti o accorpati. La norma» Il CUN con una delibera approvata ieri rivolge un pressante appello al Parlamento e al Governo perché con opportuni, ulteriori emendamenti si scongiurino i gravi rischi per la ricerca scientifica del Paese (...)» continuando. Credo allora che tutti noi, e soprattutto chi almeno all'esterno ha dichiarato gravi preoccupazioni per il mondo della ricerca, dobbiamo farci carico di tale problematica. Aggiungerò poi, Presidente, che per i regolamenti di delegificazione vi è in questo provvedimento un abuso non più tollerabile, perché vengono utilizzati al posto di deleghe legislative senza che ci siano princìpi e criteri direttivi e senza rispettare nemmeno la legge fondamentale in materia di regolamentazione da parte del Governo.

È vero, si tratta di un provvedimento complesso, che ha caratteristiche fondamentalmente fiscali, di intervento catastale, di intervento normativo su una serie di questioni. Il riconoscimento dell'urgenza e della necessità deriva dal collegamento riconosciuto di questo decreto-legge alla legge finanziaria, in quanto si tratta di uno strumento volto a dare copertura alle previsioni di entrata della legge finanziaria e questo di per sé è un elemento che motiva le ragioni dell'urgenza e dell'indifferibilità. Sapete che la legge finanziaria è già in discussione alla Camera dei deputati, in uno stato di avanzata elaborazione, ed è evidente che il decreto e la legge finanziaria si supportano a vicenda, per cui il venir meno delle norme delle norme previste da questo decreto metterebbe la legge finanziaria nella condizione di non poter essere affrontata e definita. Basterebbe questo. Ed è anche per questo motivo peraltro che, come hanno detto i relatori Benvenuto e Legnini, la maggioranza ha deciso di rinunciare all'attività emendativa su questo provvedimento. Ci si può chiedere se la prassi, instaurata da alcuni anni, di accompagnare la legge finanziaria con un decreto fiscale, anzi di anticipare la legge finanziaria con un decreto fiscale, con un decreto fiscale, sia la migliore e la più rispondente all'esigenza di mettere, da una parte il Governo, dall'altra il Parlamento, nella condizione di di definire il provvedimento finanziario, che è un provvedimento sia di bilancio annuale sia di programmazione triennale. Da questo punto di vista, è legittimo chiedersi se questa prassi instaurata da tre anni non soltanto abbia un fondamento, ma debba avere necessariamente una proiezione per il futuro. Penso che questo Governo, anche lavorando alla semplificazione e attraverso la programmazione degli interventi in materia economica e di bilancio, possa superare questa prassi dei due provvedimenti collegati - il decreto fiscale e la finanziaria - in modo da ricondurre più ordinario e più normale, quello della legge finanziaria, la programmazione annuale e pluriennale, sia per quanto riguarda le certezze che garantiscano le entrate per la finanziaria, sia avendo riguardo alla natura di un decreto fiscale, che sarebbe il caso di non caricare di temi in qualche modo ultronei rispetto allo specifico fiscale (mi riferisco alla parte alla parte che più propriamente potrebbe essere inclusa nella legge finanziaria). Ma se questa procedura diversa è auspicabile (e mi auguro che il Governo lavori a superare la prassi instaurata negli ultimi tre anni), oggi qui siamo e qui dobbiamo risolvere i problemi. Per questo ritengo che le motivazioni che hanno indotto il Governo a trattare queste materie attraverso il decreto siano assolutamente legittime e che non contrastino con la Costituzione.

di inserire nel decreto fiscale in esame una serie di normative che non hanno un immediato riferimento fiscale, pur tuttavia non credo affatto che i punti richiamati, in modo particolare dal collega Pastore, rivestano un carattere di incostituzionalità. Non capisco per quale motivo un intervento volto a definire in termini innovativi il rapporto tra concedente e concessionario in materia di autostrade debba essere ritenuto incostituzionale. Penso che sia assolutamente naturale che un sistema impositivo, ancorché ripristini in forme diverse rispetto al passato l'imposta sulle successioni, sulle successioni, trovi legittimazione nel dettato costituzionale e rientri a pieno titolo nelle facoltà di un Governo e nel potere del Parlamento di approvare o di respingere.

derivanti dalla delegificazione che, in qualche modo, potrebbero configurare - si preoccupa il collega Pastore - una sorta di abuso

anche attraverso una serie di norme ripetute nel corso dell'ultimo decennio, si sia prodotta una delegificazione probabilmente eccessiva e generica o generalista, che dà spazio all'uso del regolamento in luogo dello strumento legislativo. Allo stato delle cose, però, mi pare di capire che anche quanto richiamato nei commi 138 e 145

Signor Presidente, il decreto‑legge in esame costituisce, come sappiamo, uno dei provvedimenti cosiddetti collegati alla manovra finanziaria.

i collegati alla legge finanziaria avrebbero la funzione, visto che nella legge finanziaria non possono entrare norme ordinamentali, di occuparsi della parte ordinamentale a completamento dei valori contenuti

in funzione della legge finanziaria, che è anche decreto-legge e, quindi, introducendo delle norme di carattere ordinamentale, palesemente contraddice i criteri di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77

in oggetto comprende diversi commi che violano il disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto presentano un ambito di applicazione eccessivamente esteso e danno luogo a discriminazioni tra categorie di destinatari, precisando fattispecie di applicazione. Ma ci sono tantissimi altri aspetti all'interno di questo decreto collegato: potremmo pensare di aver stabilito una nuova figura istitutrice di norme legislative con un decreto collegato. Augurandomi

tra un decreto‑legge e la sua pseudo-urgenza e il collegato alla necessità ordinamentale di procedere), il Gruppo della Lega Nord Padania ritiene assolutamente fondata la questione pregiudiziale di costituzionalità e su questa darà il proprio voto favorevole.

Presidente, io mi rivolgerò in particolare alla sua persona, perché le chiedo la possibilità di esprimere un voto libero su questa questione e tenterò di spiegare cosa intendo per voto libero. presidente Marini, per volontà del Governo di questo Paese, noi oggi siamo all'esame delle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ieri la Commissione affari costituzionali è stata messa - e do atto di grande onestà al presidente della Commissione Bianco - nelle condizioni di non votare il parere. Oggi i membri del Governo affollano l'Aula del Senato, dopo aver negato di far conoscere il loro parere sui rilievi di costituzionalità che vedevano concordi, sia pure con sfumature diverse, maggioranza e opposizione nella 1ª Commissione. Credo Credo sia grave che i membri del Governo, che non rispondono ai rilievi della Commissione, oggi condizionino il voto dell'Aula con il loro contributo determinante. Credo anche ci sia da dire qualcosa sul merito delle questioni pregiudiziali e mi rivolgo soprattutto ai senatori a vita che sono presenti in quest'Aula. Mi rivolgo segnatamente al presidente Ciampi, alla senatrice Levi-Montalcini e al senatore Colombo: loro sono in quest'Aula perché rappresentano un pezzo importante della Nazione. Il presidente Ciampi ha servito la Nazione per sette anni e mi piacerebbe poter interloquire con lui.

riflessione ai membri della 1a Commissione affari costituzionali. Il senatore Saporito ha illustrato, a nome della Casa delle libertà, la questione pregiudiziale riferita ai 4 commi sui quali tutti abbiamo espresso perplessità. La differenza, presidente Marini, è che la maggioranza della Commissione, con il parere del relatore Villone

Chiedo ai senatori eletti all'estero: che cosa racconterete ai nostri connazionali se queste norme saranno inficiate dalla Corte costituzionale, quando anche voi doveste contribuire alla loro approvazione? Riflettiamo su un'ingiustizia che può essere commessa e che cercherò di spiegare nei pochi minuti che mi restano a disposizione.

avremmo voluto discuterne nel tempo giusto, invece accade altro. A causa dell'incapacità di ascolto della maggioranza rispetto a questo tema, promossi ricorsi da parte di quei dirigenti pubblici, nominati con contratti a scadenza pluriennale,

colleghi - che costringerà lo Stato a soccombere e comunque la Corte costituzionale a pronunciarsi, è quella subita da una persona. Presidente Marini, per la prima volta il Parlamento introduce una norma *contra personam* che riguarda il dirigente dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Costui è l'unico professionista e lavoratore autonomo

Grazie anche alla norma che consente incredibilmente di non confermare negli incarichi una persona e quindi di revocarla senza motivazioni (perché ciò è scritto nelle norme modificate dalla Camera dei deputati), sono violati l'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza di trattamento dei cittadini

con le firme dei Presidenti dei Gruppi, sicuramente sarà chiesto al Capo dello Stato un esame serio sulla costituzionalità di tali norme. Lei, Presidente, ha la carta che può aiutarci a risolvere questo problema. Abbiamo assistito già a troppi strappi io comincio ad avere, e mi dispiace doverlo dire, qualche dubbio sull'imparzialità nella conduzione dei lavori. Ci è stato impedito di discutere di tali questioni nell'esame dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione;

la questione di fiducia, posta, signor Presidente, a fronte di appena 100 emendamenti di merito su 188 commi del provvedimento (un emendamento ogni due commi). Impedisca al Governo di porre la questione di fiducia, ci faccia discutere nel merito, perché ne abbiamo diritto, perché non vogliamo approvare un provvedimento viziato da palese incostituzionalità. Questo è il motivo per cui Alleanza Nazionale sostiene convintamente sia la pregiudiziale di costituzionalità, sia la questione sospensiva avanzata dal senatore Pastore.

anche, si potrebbe dire, rendermi consapevole di un ruolo. Il ruolo del Presidente è chiarissimo, non può andare oltre ciò che deve fare.

e da me deprecata, assenza del Governo nel momento della decisione sui presupposti di costituzionalità in 1a Commissione.

l'impossibilità di porre questioni pregiudiziali su articoli ed emendamenti e in Aula oggi si è avuta la libertà di porre, come è stata posta,

che il Senato e i Gruppi nel loro lavoro creino le condizioni per poter agire evitando la fiducia. Per quanto mi riguarda, se posso, senza interferire, perché lei deve anche ricordare

colleghi, andiamo avanti con i nostri lavori.

Credo, almeno per quanto ci riguarda, che ci siamo lasciati trascinare un pochino

questo è un dato che non vuole mancare di rispetto al presidente Ciampi, ma è un fatto politico e istituzionale di gravità inaudita, perché non è possibile che una stessa persona quando è Presidente della Repubblica e deve garantire determinati criteri di costituzionalità dica «no» - e posso portare una testimonianza *pro**veritate* di ciò - e poi venga da senatore a votare provvedimenti della stessa natura in Senato. Credo che questo sia gravissimo! Senatore Castelli, io però un principio lo devo ribadire per forza: qui dentro il diritto e la libertà di voto sono assicurati a tutti coloro che sono qui, anche a titolo diverso!

non ho dato la parola alla senatrice Finocchiaro su questo problema, è inutile che continuiamo a discutere di una questione che non può trovare altra soluzione fuori da quello che ha detto il Presidente. La prego,

costituzionale e della responsabilità istituzionale che ciascuno di noi ha in quest'Aula e lei sopra tutti noi, *primus inter pares*,

Ciò detto, vorrei dire ai colleghi che stanno strumentalmente e in maniera, secondo me, poco elegante impugnando questa questione... che guardassero i numeri: anche se i senatori a vita che hanno votato con la maggioranza non avessero votato, la vostra spallata, anche stavolta, ve la siete scordata! *(Vivi, prolungati applausi

Presidente, io credo che non occorra l'intervento della collega Finocchiaro per sapere che i senatori a vita hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti noi. Non è questo ciò che noi vogliamo mettere in evidenza. Noi speravamo che i senatori a vita avessero sempre anche le stesse idee. AN)*. Questo è il problema di fondo, signor Presidente. Lei non può toglierci il diritto di protestare o, comunque, di confrontarci politicamente anche con i senatori a vita e di ricordare loro, soprattutto a coloro che hanno ricoperto la prima carica dello Stato...

abbiano gli stessi diritti e possano votare come meglio credono. Noi però abbiamo il diritto di confrontarci anche con loro e di mettere in evidenza questi atteggiamenti diversi a seconda del ruolo che ricoprono. Vorrei che questo fosse chiaro e che chiudessimo per sempre questa assurda Registriamo che i senatori a vita si sono schierati con la maggioranza; hanno il diritto di farlo; ne prendiamo atto, non ci adontiamo più di tanto. Consentite, però, a noi di poter dire quello che pensiamo sui loro atteggiamenti, singoli e complessivi.

direi che io parlo, o spero di poter parlare, a nome della categoria essendo, di quelli che volgarmente vengono chiamati "senatori pannoloni", il più giovane, quello cioè con il pannolone più piccolo. È noto che io ho sempre sostenuto che, *de* *iure condendo*, in una democrazia compiuta, che è la democrazia del più uno, in futuro, i senatori a vita debbano scomparire, i senatori di diritto debbano scomparire - l'ho detto in quest'Aula e l'ho scritto - o, come grandi consiglieri del Senato, non debbano votare. Questo *de* *iure* *condendo* ed era previsto in una delle tante riforme della Costituzione. Per esempio, era previsto dalla Bicamerale presieduta dall'amico onorevole D'Alema, dov'era prevista l'abolizione dei senatori di diritto e a vita - consentitemi - veniva dato agli ex Presidenti della Repubblica (qui siamo in tre) quello che noi non abbiamo e che è dato in tutto il mondo, cioè la pensione. Noi dovremmo formare un sindacato per chiedere la pensione In tutto il mondo i nostri colleghi hanno la pensione; pensate che il Presidente della Repubblica federale tedesca, che dura in carica cinque anni, quando va a casa mantiene lo stesso identico trattamento di quando era in carica il Presidente della Repubblica francese ha i due terzi. Ebbene, io sono dell'opinione che una democrazia compiuta è la democrazia del più uno. Quando rimproverarono a Churchill di tenersi in sella con due voti, egli rispose «Ne ho uno di più». No, era la democrazia, non era Churchill, era la democrazia che è cosa diversa! Poi, vorrei dire una cosa: in tutta la mia vita, io sono stato favorevole all'obiezione di coscienza. Quando sono stato Presidente della Repubblica ho rinviato al Parlamento la legge sull'obiezione di coscienza perché il ruolo di un Capo dello Stato e i parametri che deve usare un Capo dello Stato sono diversi e possono essere in contrasto anche con le sue opinioni politiche personali. La legge sull'obiezione di coscienza del Governo Andreotti, Governo Andreotti, che io rinviai al Parlamento il giorno prima di scioglierlo, se fossi stato deputato l'avrei votata infischiandomene dei criteri di costituzionalità; da Presidente della Repubblica l'ho rinviata al Parlamento, entrando in urto con Giulio Andreotti. Perché i criteri in base ai quali agisce un Capo dello Stato non sono criteri puramente politici, ci mancherebbe altro, anzi non debbono essere criteri politici. Se io voto e una cosa mi va, mi preoccupo assai poco. Io fui uno di quelli che, quando fu modificato il Regolamento, si batterono contro il giudizio di costituzionalità delle leggi, perché non spetta al Parlamento giudicare della costituzionalità delle leggi e questa è una cosa che - mi dispiace - vollero gli amici di sinistra per mettere altri ostacoli alla maggioranza di allora. Quindi, che un Presidente della Repubblica abbia votato qui politicamente in modo difforme da quello in cui ha preso alcune decisioni come Capo dello Stato,

*(UDC)*. Signor Presidente, ho molto apprezzato l'intervento del senatore Cossiga, dal quale mi permetto di dissentire su due punti. Il primo questo riferimento vagamente iettatorio alla scomparsa dei senatori a vita; lunga vita ai senatori a vita, almeno empiricamente, come categoria giuridica poi vediamo. Il secondo punto è che non credo che il Parlamento possa infischiarsene dei criteri di costituzionalità. Non credo che un deputato, chiamato a rappresentare il popolo italiano sulla base della Costituzione vigente, possa votare

il vincolo costituzionale, quando avremo una Costituzione non rigida come l'attuale, ma elastica, variabile, non scritta, liberamente sfondabile da qualunque prevaricazione parlamentare, lei avrà ragione. Tuttavia, finché vige la Costituzione attuale, sulla base di essa, i parlamentari quando votano un giudizio di costituzionalità devono occuparsi non del vantaggio politico della loro ma dell'effettiva costituzionalità del provvedimento. Sarebbe pericoloso far passare il principio da lei enunciato, anche se ha avuto gli applausi - per la verità fiacchi - della maggioranza. Vorrei poi mettere in evidenza un'altra questione. Certo, la Costituzione vigente è una cosa, quella futura e sperata è un'altra, tuttavia, sarei esitante nel dire che un senatore a vita è un senatore come tutti gli altri. Certo, egli ha gli stessi diritti di tutti gli altri ma, forse, ha qualche dovere in più. Io non metto in questione che i senatori a vita votino secondo coscienza. Ma anche solo fornire il dubbio

ma quelle di opportunità politica; anche solo fornire il dubbio di non sentire quel dovere di imparzialità da loro onorato con altissime cariche e, quindi, il dovere di essere al di sopra della polemica politica contingente

per elevare il tono del confronto parlamentare e fare in modo che in tutti prevalga la preoccupazione per il bene del Paese sulla preoccupazione di parte e sulle discipline di coalizione e di partito. *(Applausi

mi permetto di avanzare una proposta per uscire da questa polemica che si ripete periodicamente. Ponga all'ordine del giorno del Senato il disegno di legge presentato dal senatore Cossiga in merito alle prerogative e ai diritti dei senatori a vita. Discutiamone, con l'impegno dei senatori a vita a non partecipare alla votazione su tale disegno di legge. Se il Senato, attraverso la procedura parlamentare di approvazione di una legge di ordine costituzionale

prospettare l'ipotesi - e la maggioranza purtroppo lo fa - di avere l'arma di riserva nei senatori a vita, allora si cancella tutto il discorso di natura istituzionale e delle prerogative e dei diritti dei senatori a vita, che nessuno di noi vuole discutere.

Esercitino i loro diritti, ma rispondendone personalmente con la loro presenza, il loro voto e la loro faccia. E' inaccettabile una sostituzione, quella sì su base politica e di appartenenza alla coalizione, che a loro non compete.

Lo avevo intuito e mi congratulo per la straordinaria comunità di pensiero che il suo Gruppo dimostra, perché, alla fine, il senatore Stracquadanio ha detto ciò che lei ha rafforzato.

che al Senato la maggioranza di senatori non corrisponde alla maggioranza elettorale nel Paese, che vi ha visto soccombenti per 250.000 voti. Il mio intervento sarà di natura regolamentare, Presidente. Non vi è dubbio che la Costituzione attribuisca il diritto di esprimere il voto anche ai senatori a vita.

Ve ne sono due che normalmente frequentano l'Assemblea e le Commissioni... delle fiducie o quando cade il Governo, no! Vadano a lavorare, perché prendono lo stipendio come tutti gli altri e rendano onore all'articolo 1 del nostro Regolamento!

a questa sgrammaticatura istituzionale che offende noi stessi, nel momento stesso in cui offende il ruolo e la funzione dei senatori a vita, passando al merito del problema e

Allora, mettiamoci d'accordo su due punti fondamentali, perché la Costituzione dovrebbe reggere i nostri lavori. Mentre diciamo, come altri Gruppi di maggioranza ed altre senatrici e senatori, grazie per la funzione che hanno svolto

quali è che la differenza tra le senatrici ed i senatori eletti ed i senatori e le senatrici a vita è semplicemente, costituzionalmente, nel modo in cui si è formata la rappresentanza, ma il *collegium* (il collegio) è nella sua interezza, con pari diritti e pari doveri. Questo lo insegniamo al primo anno di università ai nostri studenti, non voglio insegnarlo qui - non mi permetterei mai di farlo - ad autorevoli esponenti dell'opposizione.

funzione costituzionale. Non c'è dubbio su questo punto e io credo che abbiamo prodotto delle pesanti sgrammaticature istituzionali questa mattina, di cui mi scuso con le senatrici ed i senatori a vita, perché, come diceva il saggio della mitologia: «Iddio acceca chi non vuol vedere». Veramente Iddio acceca chi non vuol vedere. Io credo vi sia un problema politico relativo a tale accecamento. Il problema politico è che si era favoleggiato tanto

perchè non vogliamo la fiducia, vogliamo il confronto in Parlamento e lo vorremo per tutta la prossima settimana. Voi avete una difficoltà politica. Non a caso, non vedo oggi nelle tribune il cavalier Berlusconi, che aveva promesso di essere qui ma forse ha capito che andava al massacro e non è venuto; forse siamo alla barbarie che voi avete dimostrato contro i senatori a vita, perché, quando un impero crolla, anche la barbarie viene fuori.

per chi parla non vi è mai stato dubbio che i senatori abbiano tutti pari dignità istituzionale e costituzionale. però anche pari dignità politica sia nel dare consigli, suggerimenti ed esprimere il loro voto, sia nel ricevere critiche e valutazioni che incidono sugli atteggiamenti che tengono in Aula o eventualmente nelle Commissioni, laddove siano presenti in quella sede. Credo che abbiamo non solo il diritto, come diceva il collega Matteoli, il dovere di rappresentare agli italiani le incongruenze, le contraddizioni e gli atteggiamenti ambigui di tutti i senatori, anche, credo che nessuno possa negarlo, dei senatori a vita,

che l'intero Paese ha sentito come propri rappresentanti, e che oggi sono platealmente schierati da una parte, cioè rappresentano metà del Paese. Signor Presidente, credo sia allora doveroso per noi, come possiamo fare per qualsiasi senatore, che magari su argomenti particolari nella sua vita accademica, professionale, imprenditoriale e giornalistica, ha espresso delle opinioni, contestare le contraddizioni e le incoerenze con le opinioni espresse;

quando si è fuori da quest'Aula e poi impunemente, cioè senza critiche, pensare di sostenere una tesi opposta dentro quest'Aula. Noi che siamo eletti dal popolo abbiamo grandissime difficoltà e grandissimi tormenti quando dobbiamo, magari per disciplina di partito, assumere atteggiamenti che contrastano con le nostre prese di posizioni passate:

di diritto o scelti dal Capo dello Stato - non abbiano avvertito un sussulto di dubbio sulla legittimità di questa norma, che viene contestata

atteggia a vestale, a nume, a tutrice della ricerca e poi vota a favore di questo provvedimento, di una norma palesemente incostituzionale sul tema della ricerca: abbiamo il dovere, l'obbligo, oltre che il diritto, di evidenziare questo dato e di contestarlo. Quindi credo che oggi si chiariscano i punti della discussione: nessuna contestazione sul piano istituzionale, ma una chiara conferma che i senatori a vita, o la gran maggioranza di loro, sono schierati con il centro-sinistra, non solo per le grandi scelte, come possono essere quelle istituzionali, ma anche per il cammino naturale e normale di quest'Aula e questo mi sembra molto grave sul piano politico e forse anche sul piano etico.

all'attenzione di tutta l'Aula. Sono d'accordo con quanto espresso dal presidente Calderoli nel suo intervento, nel senso che noi abbiamo assunto, da un po' di tempo, l'abitudine di sottolineare con applausi o altre manifestazioni qualunque risultato su qualsiasi decisione: credo sia un errore *bipartisan*,

ton* proprio della Camera alta, del Senato della Repubblica. Le decisioni sono tali, in un percorso complessivo, e sono tante: se ad ogni decisione c'è una sottolineatura

Mi pare che se adottassimo provvedimenti regolamentari o legislativi sulla base di un momento di forti passioni, potremmo commettere qualche errore. Concludo dicendo che a noi serve altro, invece: serve recuperare quella scioltezza e quell'eleganza proprie del Senato della Repubblica e serve a tutto il Senato fare in modo che i nostri senatori a vita, *de iure condito*, continuino a mantenere, insieme al bagaglio di esperienza che possono portare, la loro autonomia di giudizio e di pensiero. Credo che questo sia ciò che più ci debba stare a cuore: avere dei senatori a vita che, per quello che hanno rappresentato per la Nazione, possano portare in autonomia di giudizio e di pensiero

perché sentire grida e contestazioni così forti nei confronti di una delle donne più prestigiose che abbiamo in Italia, come Rita Levi-Montalcini, di un presidente amatissimo dagli italiani, come il presidente Ciampi, o di un presidente prestigioso, come il presidente

Ciò mi pare del tutto elementare e quindi è inutile che ci si torni sopra. Credo che sia successa un'altra cosa e vorrei sottolinearlo. E' accaduto che, anche ad opera di quei giornalisti che vengono chiamati retroscenisti, parecchi in Aula si aspettavano una qualche sorpresa. Invece è successa un'altra cosa. È accaduto che la maggioranza ha dimostrato di essere compatta. di essere forte, di farcela al di là dei senatori a vita e siete stati così delusi da un'attesa che avevate incamerato, quella di cui avevano scritto questi nostri giornalisti prestigiosi,

l'attenzione dell'Aula su un argomento che credo stia a cuore a tutti. Mi riferisco alla situazione che si sta sviluppando in Libano nella fascia affidata anche al controllo dei nostri uomini. Venerdì 6 ottobre il corrispondente dal Libano, Toni Capuozzo, nell'articolo «Hezbollah fa arrivare camion di missili e UNIFIL osserva», pubblicato sul quotidiano «Il Foglio», denunciava la rioccupazione, da parte di formazioni militari di Hezbollah, delle posizioni nell'area compresa tra il Litani e il confine israelo-libanese. da tali posizioni Hezbollah aveva lanciato i suoi missili contro Israele. Immediatamente, con una mia dichiarazione ripresa dagli organi di informazione, avevo chiesto conferma

il Governo libanese ha segnalato all'inviato per il Medio Oriente dell'ONU, Terje Roed-Larsen, che le infiltrazioni di armi provenivano impunemente dalla Siria a favore di Hezbollah. I dirigenti di Beirut hanno sottolineato che il traffico continua, nonostante la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza, attraverso la quale si pone l'embargo a tutte le armi destinate al «Partito di Dio».

il senatore Ramponi ha ragione. Pregherei i colleghi di prestare grande attenzione. Non confondiamo l'attenzione con la presenza, sono due cose diverse. Pregherei i colleghi presenti nell'emiciclo di prendere posto o accomodarsi fuori, altrimenti è difficile parlare, soprattutto quando si trattano argomenti così importanti. RAMPONI *(AN)*. Dal canto suo, la Siria aveva risposto che era probabilmente in atto un traffico di armi dalla sua frontiera verso il Libano, precisando che il confine è difficile da sorvegliare.

«Temiamo che la situazione possa deteriorarsi rapidamente nella zona e in molti modi, in particolare con azioni che potrebbero essere avviate a partire da questa zona in direzione di Israele». Da parte loro, i servizi di sicurezza israeliani hanno annunciato che Hezbollah si sarebbe rinforzato militarmente e disporrebbe oggi di ben 20.000 testate di missili. A questo punto, ritengo sia davvero irresponsabile da parte del nostro Governo continuare ad ignorare una situazione che nei suoi sviluppi conferma quello che annunciò Toni Capuozzo un mese fa e che trova ripetute conferme. È impossibile ignorare il deterioramento della situazione e, a mio parere, è irresponsabile non informare il Parlamento di una situazione che riguarda più di 2.000 nostri uomini: informarlo nei termini in cui fu promesso al momento in cui, tutti assieme, concordi, decidemmo di inviare il nostro contingente per assicurare la tregua. È irresponsabile, specie nei confronti dei nostri soldati che, come dicevo, abbiamo inviato tutti assieme, senza dare loro, come abbiamo ripetutamente denunciato, chiare indicazioni su quelli che chiamiamo

i nostri lavori perché il senatore Ramponi sta parlando di argomenti importanti, che riguardano i nostri militari all'estero, in missione.

che il Governo venga tempestivamente a riferire, qui in Senato, sulla reale situazione nella quale vivono i nostri soldati

suoi motivi di preoccupazione vorrei aggiungere quanto sappiamo bene - per averlo letto sui giornali - e cioè che tre giorni fa il presidente dell'Iran, Ahmadinejad, ha detto che presto Israele sarà cancellato e distrutto dalle carte geografiche. Prima l'aveva auspicato, adesso l'ha messo in forma di previsione. Si sa anche - ma è meno noto - che il 19 ottobre lo stesso generale Pellegrini, comandante dell'UNIFIL e dunque anche dei nostri soldati in Libano, ha auspicato di poter usare non solo mezzi diplomatici per contrastare i sorvoli fatti da Israele sul Libano, pur sapendo (le fonti che hanno reso noto la notizia ne hanno altresì reso conto) che questi sorvoli questi sorvoli vengono fatti per impedire che quanto meno le armi arrivino agli Hezbollah dall'Iran per via aerea. Quindi, mettendo insieme le dichiarazioni di Ahmadinejad, che prevede una una pronta scomparsa dello Stato di Israele, alla situazione descritta dal senatore Ramponi si dovrebbe indurre il Governo a venire a riferire spontaneamente, anche perché il 18 agosto nelle Commissioni esteri e difesa riunite di Camera e Senato

quale ha affermato che ogni problema dell'area deriva da Israele. Questo non ci rassicura per nulla né sulla dignità della nostra posizione sul piano internazionale, né tanto meno sulla sicurezza dei nostri soldati che si trovano in Libano su mandato dell'ONU e su mandato di questa Camera.

e Malan. Vorrei chiederle se stiamo aprendo un dibattito sulle questioni relative alla missione italiana o, meglio, alla missione UNIFIL delle Nazioni Unite in Libano, al suo esplicarsi,

Se vogliamo aprire un dibattito tra tutti i Gruppi sul tema, vorrei ricordare a chi mi ha preceduto che la Commissione difesa ha già chiesto al Ministero di fare un sopralluogo in Libano, che la Commissione difesa, nell'ambito di un'indagine conoscitiva, proprio pochi giorni fa (il collega Ramponi lo sa bene), ha tenuto un incontro nel palazzo delle Nazioni Unite con la cellula che sovrintende alla gestione della missione UNIFIL e che in quell'occasione la Commissione difesa, rappresentando il Senato della Repubblica, ha avuto la possibilità di uno scambio di informazioni e di comunicazioni, con quella stessa cellula, relativamente al sorvolo degli aerei israeliani in quell'area e alle preoccupazioni dell'eventuale passaggio di armi. Tuttavia,

Lei sa, senatore Nieddu, che ci sono tecniche parlamentari e regolamentari che consentirebbero a chiunque di prendere la parola e non finirla più.

non entrando nel merito delle dichiarazioni del senatore Ramponi, le richiamo, ritenendo che sia utile che il Governo venga a riferire in Aula sulla situazione che si sta determinando in Libano.

portare al compendio di alcune notizie utili all'intero Senato. Mi associo dunque alla richiesta del senatore Ramponi.

alla risoluzione delle Nazioni Unite 1701, i Governi degli Stati membri sono chiamati al rispetto della risoluzione 1559 dell'ONU, che

alla posizione assurdamente equidistante che ha tenuto fino adesso.

Si tratta della trasposizione in un emendamento e in un ordine del giorno del parere espresso dalla Commissione finanze del Senato sul provvedimento al nostro esame.

di un nuovo sistema multilaterale di negoziazione. Cosa vuol dire? Con la legge comunitaria stiamo recependo una delle direttive in materia finanziaria più importanti nella storia dell'Unione, quella che cambia l'infrastruttura del sistema finanziario europeo e quindi, probabilmente, anche la struttura. In particolare, viene superato il meccanismo di obbligo di concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati attraverso, per l'appunto, la possibilità di predisposizione di sistemi multilaterali di negoziazione di sistemi multilaterali di negoziazione - chiamiamoli propriamente privati - che rendono possibile, in quanto in concorrenza tra di loro, di abbassare i prezzi delle negoziazioni dei titoli finanziari. Perché è importante quello che ieri annunciava la stampa finanziaria internazionale? Quelle sette grandi banche, che realizzano un nuovo sistema multilaterale di negoziazione, rappresentano più o meno la metà del complesso delle negoziazioni sui mercati finanziari europei.

C'è il rischio, cioè, che nel nuovo quadro, che modifica complessivamente i mercati finanziari europei, l'Italia accumuli ritardi; quindi, è importante provvedere a recepire la direttiva. In particolare, richiamo l'attenzione del Ministro su una delle proposte contenute all'interno dell'ordine del giorno Come vengono disciplinati i sistemi multilaterali di negoziazione? C'è una direttiva e ci sono alcuni regolamenti molto dettagliati dell'Unione Europea. Come rendiamo possibile, per i soggetti italiani, predisporre queste piattaforme e questi sistemi?

Per dirla brutalmente, chi vuole predisporre questi sistemi, visto il dettaglio delle norme già previste, può semplicemente fare uno statuto che rispetti quelle norme e l'autorità di vigilanza si adeguerà.

Così com'è formulato, il testo al nostro esame prevede che questa rischiosità debba essere individuata titolo per titolo. Sembra un provvedimento più rispettoso della tutela dei risparmiatori; in realtà non lo è.

noi abbiamo difeso in Commissione, ha trovato una soluzione eccellente, anche per lo sforzo del presidente Manzella e del presidente Benvenuto; diamo atto della soluzione individuata, che consente

anche su sollecitazione del Governo, che facessero prevalere le società di capitali. Con le opportune garanzie, si tratta di una soluzione intelligente. Detto questo, dichiaro di

perché riteniamo che non si debba stare sotto indicazioni generiche, ma si debba attentamente valutare la rischiosità dei prodotti. Detto ciò, Presidente, credo che questa legge comunitaria, per la quale siamo impegnati in una pronta approvazione, contiene scelte forti, come quelle appunto contenute all'articolo 10, che recepiscono la cosiddetta direttiva MIFID che è una pietra angolare sul piano di azione per i servizi finanziari, per l'affermazione di un mercato unico europeo e una risposta ai mutamenti strutturali sul mercato dei valori mobiliari. Vengono poste regole chiare e prevedibili per offrire maggiore sicurezza agli investitori e ai consumatori che acquistano servizi da imprese estere e questa direttiva avrà un ruolo essenziale per realizzare un mercato dei capitali più integrato, più efficiente, per ridurre i costi del capitale e favorire la crescita nella competitività. Prima approviamo queste norme e prima interverrà l'adeguamento successivo. È una sfida per il Paese che vuole misurarsi con nuove sfide - quelle che ricordava prima il senatore D'Amico - delle piattaforme tecnologiche rispetto alla quale il Paese non può rimanere in una posizione subordinata e le banche saranno chiamate a nuove sfide, con nuovi investimenti. Diciamo subito, però, onorevole D'Amico, che non c'è piaciuta la scelta di abrogare gli articoli 9, 10 e 14 della legge sul risparmio attraverso la legge comunitaria; una scelta improvvida! Non c'è piaciuto il mancato esercizio della delega non c'è piaciuto che prevalgano *lobby* in questo Governo, come quanto è accaduto alla Camera dove hanno risposto a un preciso disegno politico rispetto all'articolo rispetto all'articolo relativo al 30 per cento, alla sterilizzazione dei diritti di voto per le fondazioni bancarie. Non c'è piaciuto che il vice ministro Pinza abbia operato una controriforma con un parere asimmetrico rispetto a quello che abbiamo approvato in Senato, attraverso un parere su un decreto legislativo su un argomento chiaramente fuori delega. È per questo che abbiamo, signor Presidente, apprezzato la misura del presidente Benvenuto che è stato rispettoso delle regole e ha impedito questo parere così asimmetrico. Dico subito, Presidente, che non ci può essere un conflitto di interessi soltanto quando parliamo del presidente Berlusconi; in questo parere, espresso dalla Camera, c'è stato un chiaro

perché riteniamo che i consumatori debbano essere tutelati con indicazioni precise. È stato risolto felicemente, come ho detto, il problema dei consulenti finanziari indipendenti. Non è solo aver evitato uno stravolgimento della direttiva rispetto al principio di libertà, che è quello di esercitare una professione non solo in forma di società, ma anche con le opportune garanzie, anche in forma individuale. Molto opportunamente, Presidente, non è stata calata in questa legge comunitaria la direttiva sull'OPA, anche grazie all'intervento del senatore Buttiglione, richiedendo maggiore attenzione da parte del Parlamento nell'affermazione di princìpi e nell'esaltazione del ruolo, quello parlamentare, non solo nella fase ascendente, ma anche in quella discendente della normativa comunitaria. Questa è stata una scelta rispettosa del Parlamento ed è stata la nostra reazione ad impedire un esame frettoloso, senza opportuni approfondimenti rispetto a tematiche complesse che riguardano la difesa degli interessi nazionali, il principio di reciprocità e l'apertura dei mercati. Scelte difficili, che non possono appartenere ad oscure OPA manageriali senza piano industriale, come quella vista in vista in questi giorni. Per queste ragioni, signor Presidente, esprimiamo voto favorevole su questo articolo importante, nello spirito europeista che contraddistingue la nostra storia politica e parlamentare.

riguarda le attività di consulenza e la figura dell'esercente individuale di tali attività. Essendo stato recepito in Commissione, lo ritiro.

10.14, il Governo concorda con l'esigenza che gli obblighi di informazione ai consumatori siano fatti per tutti gli strumenti finanziari. E' un dato importante e in questo senso il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

e 10.29 il parere è contrario. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G10.100, di contenuto molto vincolante, come il proponente certamente sa, il Governo lo accetta come raccomandazione.

che l'ordine del giorno G10.100, pur meritevole nelle sue indicazioni, è una forma edulcorata del parere che lo stesso senatore D'Amico aveva espresso in Commissione finanze. Ritengo sarebbe stato più utile recepire le intere indicazioni formulate nel parere. Non possiamo scegliere questa strada così edulcorata che troveremo nuovamente quando affronteremo il problema del decreto fiscale e della legge finanziaria, cioè risolvendo i problemi attraverso gli ordini del giorno.

l'opposizione e parti della maggioranza per salvaguardare nel nostro ordinamento la figura del consulente finanziario, lasciando anche alla libera professione la possibilità di esercitare questo compito senza vedere, nell'assegnazione solo a banche o solo a SPA, ridotta una quota di mercato e sottratta a quel processo di liberalizzazione al quale noi invece tutti puntiamo. Siamo contenti di aver trovato nel ministro Bonino ed in parti di questa maggioranza, come quella rappresentata dal senatore Silvestri, la nostra stessa sensibilità.

Benin: reclusione da uno a tre anni più un'ammenda; Bhutan: fino alla reclusione a vita; Botswana: reclusione per un periodo non inferiore a sette anni; Brunei: reclusione fino a dieci anni e un'ammenda; Burma/Myanmar: reclusione fino ad un anno; Burundi: l'omosessualità è punita come atto immorale; Cayman: reclusione; Camerun: reclusione da sei mesi a cinque anni più un'ammenda; Capo Verde: reclusione da stabilirsi per rapporti contro natura e contro la decenza pubblica e personale; Cina (di cui parleremo oggi pomeriggio): reclusione fino a cinque anni, anche se non c'è un articolo esattamente antiomosessualità; Isole Cook (protettorato Nuova Zelanda): reclusione fino a sette anni; Cuba: reclusione da tre mesi ad un anno per la manifestazione pubblica di omosessualità; Gibuti: reclusione con durata da stabilirsi; Egitto: reclusione o lavori forzati fino a cinque anni; Emirati Arabi Uniti: per alcuni emirati fino a sette anni di reclusione; Etiopia: reclusione da dieci giorni fino a tre anni; Fiji: reclusione fino a quattordici anni; Gambia: reclusione fino a quattordici anni; Giamaica: reclusione e lavori forzati fino a dieci anni; Ghana: reclusione da stabilirsi, ma vi sono anche testimonianze di torture; Grenada: è illegale ma non si hanno notizie di pene; Guyana: reclusione fino a due anni; Guinea: reclusione da sei mesi fino a tre anni e un'ammenda; India (con la popolazione che ha): reclusione a vita; Iran: pena di morte (se minorenne, cento frustate);

Libano: reclusione fino a un anno; Liberia: reclusione per un periodo da determinarsi in base alla volontarietà; Libia: reclusione da tre a cinque anni; Liberia: reclusione fino a tre anni; Malawi: reclusione, ma il cittadino occidentale è salvaguardato; Malesia: reclusione da due a vent'anni; Maldive: reclusione; Mauritania: pena di morte; Marshall: reclusione fino a dieci anni; Mauritius: reclusione fino a cinque anni; Marocco: reclusione da 6 mesi a cinque anni; Mozambico: reclusione fino a tre anni; in Namibia non è tollerata ma non vi sono leggi contrarie; Nepal: reclusione; Nicaragua: reclusione fino a tre anni;

Sierra Leone: non si hanno notizie di reclusioni; Singapore: reclusione a vita; Siria: reclusione fino ad un anno; Isole Salomone: reclusione fino a quattordici anni; Somalia: reclusione da tre mesi a tre anni;

Cari colleghi, ho voluto leggervi questa lunga lista per chiarire che ciò che stiamo votando non è una questione ideologica, non c'entra alcunché con i PACS, con la famiglia, con le convinzioni personali di chiunque, è una norma di civiltà che può salvare la vita a molte persone che nel loro Paese rischiano la pena di morte o lunghissime pene detentive. Voglio anche

a tutti rispetto a tali questioni. Purtroppo, per poter accedere a tale questione ci vuole una coscienza individuale che solo la democrazia, le società civili avanzate e un forte movimento consentono di avere: quelli che chiederanno asilo saranno proprio gli oppressi, non certo gruppi auto-organizzati, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di tale norma. Chiudo usando le bellissime parole di Franco Fortini: «Molte volte la sessualità è stata luogo ove una folla tace e gli amici non riconoscono». Non vi chiedo di riconoscere questo, ma di riconoscere il diritto

perché non c'entravano nulla con gli internati fascisti, di aprire finalmente orizzonti in cui tutti abbiano la possibilità di vivere.

comunque gli strumenti per esercitare il proprio diritto alla difesa. Una sola notazione: nella discussione generale tutti i colleghi hanno introdotto l'esigenza di rendere più cogente il ruolo del Parlamento anche nella fase discendente. non è lo strumento più adatto, ma comprendiamo tutti ed accettiamo questo criterio in funzione dell'esigenza di abbreviare i tempi per evitare un ulteriore numero di infrazioni. Questo però fa sì che la delega non sia

in funzione dell'espressione compiuta del ruolo del Parlamento nell'indirizzo della delega al Governo, proprio per accrescere, anche con l'utilizzazione di questo specifico strumento, la partecipazione all'Assemblea elettiva, così come rivendicata da tutti i Gruppi. *(Applausi

introdotto l'articolo 12, ossia il contenuto che a questo punto è diventato l'articolo 12. Il ministro Bonino - così mi risulta dalla lettura del Resoconto - ha chiesto di non inserirlo o quantomeno si è rimessa all'Assemblea, per cui ha

Tale richiamo non costituiva in nessun modo un criterio di esercizio della delega, uno di quei criteri che sono obbligatori per Costituzione: l'articolo 76 della Carta fondamentale dichiara chiaramente che il Governo può agire per delega solo sulla base di criteri e tempi precisi. La menzione dell'articolo 10 non costituiva alcun criterio. è stato soppresso anche per l'ineleganza della citazione, perché è del tutto superfluo specificare che il Governo deve rispettare la Costituzione nell'esercitare una delega. Da ciò però deriva che, anziché avere un cattivo criterio, vago e forse addirittura fuorviante, adesso non abbiamo alcun criterio. Il Governo ha, infatti, una delega in bianco nel decidere esattamente quello che vuole per l'attuazione di di questa direttiva dell'Unione Europea, sulla quale non c'è nessun pericolo, né imminenza di infrazione, perché essa impegna gli Stati ad uniformarsi soltanto dal 1° dicembre 2007 e, per l'articolo 15, soltanto dal 1° dicembre 2008; non c'è quindi nessuna fretta, da questo punto di vista. Aggiungo anche che tutti i Gruppi dell'opposizione alla Camera, sul complesso del provvedimento, a causa di questo articolo, si sono espressi o con il voto contrario o con il voto di astensione.

con l'impegno nei confronti dei Gruppi dell'opposizione a discutere in tempi brevi una legge che garantisca e regolamenti in modo adeguato ai tempi, e naturalmente alla Costituzione, il diritto d'asilo. Ricordo che proprio l'articolo 10 della Costituzione, che prevede il diritto all'asilo in determinate circostanze, prevede altresì che esso sia regolamentato dalla legge, non da un decreto legislativo. Tale richiamo

stabilisce che i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere nello Stato membro ai fini esclusivi della procedura fintanto che l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo procedure di cui al capo terzo, eccetera.

Allora, la forma più coerente, che il Governo sicuramente eserciterà (è inutile nascondercelo), sarà quella di dare semplicemente la libertà di stare nel territorio italiano: quando il giudizio arriverà, le persone

legge sull'immigrazione; la maggioranza ha tutti i diritti di cambiarla, se lo ritiene opportuno (ce l'ha scritto nel programma con il quale si è presentata davanti agli elettori), ma non ha il diritto di farlo aggirando la legge: non si può cambiare una legge attraverso un decreto legislativo che tratta, in apparenza, di un altro argomento. Se in questo Paese chiunque può arrivare e chiedere diritto di asilo e, dunque, ottenere il diritto a restare per un certo tempo per poi rendersi irreperibile, allora ogni limite all'immigrazione diventa veramente superfluo. Sarebbe più logico dire, come ha fatto

che il Governo avrà emanato il decreto legislativo relativo a questo articolo, sarà possibile entrare nel nostro Paese: basta volerlo fare e basta chiedere l'asilo politico sulla base di qualunque pretesto. Perché

il Governo Berlusconi non ha mai tentato di introdurre nella legge comunitaria delle riforme su argomenti delicati e importanti e sui quali c'è la nostra disponibilità a discutere, come quello del diritto di asilo. Ribadendo

con i tempi adeguati e rispettando la Costituzione, la quale chiede che il diritto di asilo sia regolamentato dalla legge, non da un decreto legislativo fatto su carta bianca, in violazione anche dell'articolo 76 della Costituzione!

questo non è quanto ci chiede l'Unione Europea e quindi su questo bisogna essere straordinariamente precisi e puntuali. Vorrei svolgere qualche considerazione

aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Tra i gravi motivi sono inclusi quelli relativi alla discriminazione e alla repressione di comportamenti non considerati come reato dalle leggi italiane"». Non è infatti possibile andare dietro ad una elencazione che è comunque insufficiente, che lascia fuori alcuni comportamenti e che privilegia alcuni tipi di comportamento a danno di altri. Non mi nascondo che questo sarebbe un atto di grande generosità della Nazione italiana, perché ovviamente ci renderebbe recipienti di flussi di rifugiati particolarmente robusti. Sarebbe, però, un atto di grande civiltà con il quale io sarei d'accordo,

Presidente, intervengo anch'io sulla questione toccata dal senatore Buttiglione. Credo che il senatore Silvestri abbia posto una questione vera.

poi ho ascoltato, perché il dibattito parlamentare serve soprattutto a questo (lo vorrei dire ai colleghi che troppo spesso dimenticano di ascoltarsi),

fronte al dubbio che si aveva alla lettura dell'emendamento, il dibattito ci è servito a capire che si entra anche nella sfera dei diritti e della dignità della persona. Di questo stiamo parlando.

anche accogliendo la riformulazione proposta dal collega Buttiglione. Porta a casa il risultato della grande sensibilità che entra in una legge del Parlamento attorno a una questione che lui ha avuto il merito di sollevare e che nessuno può sottovalutare.

Signor Presidente, credo che occorra fare un minimo di chiarezza sui temi che stiamo affrontando, perché, pur

Vorrei ricordare che la direttiva comunitaria (della quale l'articolo 12 vuol rappresentare un'attuazione, ancorché estremamente stringata) riguarda le procedure minime per riconoscere lo stato di rifugiato. Ebbene, lo stato di rifugiato è definito da una convenzione internazionale, perciò due sono le conseguenze che potrebbero derivare da emendamenti di sostanza: l'una, che quel caso già sia previsto nella convenzione internazionale e, quindi, sarebbe norma superflua; oppure che quel caso sia al di fuori della convenzione internazionale e noi apriremmo, senza una valutazione di carattere politico

correremmo il rischio di determinare una situazione di scompenso nell'ambito comunitario. Badate, colleghi, il caso prospettato fa riflettere,

esteriori, estetici o sociali, sono ritenuti da altri Stati come reati; non vedo perché, applicando la stessa logica, anche questi comportamenti non debbano essere attratti dall'emendamento del collega Silvestri. una grande attenzione, ritenendo personalmente che si tratti di ipotesi disciplinate da una normativa internazionale alla quale si rifà la direttiva comunitaria e che questo Parlamento, anche volendo, non può modificare, né in peggio, né in meglio. Il discorso poi è assolutamente aperto sul piano

l'elenco della colonna infame di quei Paesi nei quali le convinzioni personali, le propensioni sessuali e il modo di vivere di ciascuno sono considerati delitto. Confondere il diritto con il delitto è una delle cose peggiori che possa succedere nel mondo. Ho ascoltato, inoltre, con altrettanto rispetto, il consiglio, il parere e l'opinione che ha espresso il senatore Buttiglione. Anche questo è un elemento che mi fa piacere cogliere in quest'Assemblea, dove spesso i fattori emotivi e passionali prevalgono su quelli razionali e in cui le logiche di schieramento sono spesso foriere di un atteggiamento manicheo, manicheo, preventivo e presuntivo di buone ragioni e che, secondo me, non dovrebbero essere sempre accolte. Il collega Silvestri ha posto un problema vero, un problema umano che riguarda l'intimità di ciascuno nel quale si intromette lo Stato, o meglio, gli Stati che ritengono di censurare un comportamento rimesso alla libera scelta di ciascuno di noi, o di loro, Buttiglione ha fatto una proposta che si inquadra anche sul piano giuridico, per evitare, come dicevamo prima confidenzialmente con la ministro Bonino, che un caso specifico

hanno già detto in molti, e in particolare il senatore Storace, riassumerò la nostra posizione con una, se volete, apodittica definizione, vale a dire che l'indicazione di un reato potrebbe escludere invece la generalità dei reati per la concessione dell'asilo politico ad altri.

per precisare un aspetto, in dissenso rispetto all'opinione espressa dal collega Pastore. Le convenzioni internazionali in materia di asilo ai rifugiati, così come tutte le convenzioni sui diritti umani, prevedono degli *standard* minimi ai quali ciascun Paese, per il solo fatto della sottoscrizione, è obbligato. Nessun Paese può andare al di sotto di quegli *standard*, ma addirittura tali convenzioni prevedono e auspicano che ciascun Paese sottoscrittore adotti misure più avanzate rispetto a quelle previste dalle convenzioni.

"Tra i gravi motivi sono inclusi quelli relativi alla repressione penale di fatti non previsti come reato dall'ordinamento italiano"».

che dal nostro punto di vista allude allo Stato di diritto e anche all'identità della civiltà giuridica del nostro Paese. Non comprendo perché un testo che conteneva il riferimento al terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, cioè

rimanda ad un problema di gerarchia delle fonti che è molto importante e che ha già discusso, nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati quando si è trattato - e la Ministro lo ricorderà - del mandato di arresto europeo.

che è concesso l'asilo allo «straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana». Questo è un punto qualificante non della Costituzione (o di quel che c'è) di Riyadh, di Islamabad, di Lagos o anche di Varsavia, ma della Costituzione italiana. Chi legge i lavori preparatori della Costituente sa benissimo che questo tema è stato discusso; i nostri costituenti hanno voluto salvaguardare i diritti, le opinioni, le libertà - io sono d'accordo con il senatore Buttiglione: va allargato anche a quelli che non sono considerati reati - che la nostra Costituzione e il nostro Stato di diritto prevedono per ogni donna e per ogni uomo, non, appunto quelli di Lagos, di Islamabad o di Riyadh. Questo è un tema fondamentale, che, nel momento in cui stiamo costruendo, *ex* articolo 56, la legge sull'asilo, deve improntare l'identità di uno Stato. Credo, quindi, il compromesso, o comunque l'accettazione dell'abrogazione della lettera *a)*, sia un peggioramento, nella civiltà giuridica, dello stesso diritto d'asilo. Io la penso così; per quanto mi riguarda vorrei che su questo si aprisse un dibattito vero, costituzionale. La Costituzione non è - mi permetta, Ministro - da discutere in termini politicisti; la Costituzione per me è ancora un testo sacro. Questo dice la Costituzione. Io non voterò,

dal precedente Governo, si sono voluti inserire alcuni punti del tutto incompatibili con la stessa normativa comunitaria, unicamente su pressioni di una certa sinistra, che ha messo in difficoltà la stessa ministro Bonino. Sopprimendo l'articolo 12, noi permettiamo semplicemente di recepire la direttiva del Consiglio n. 85 del 1° dicembre 2005 così com'è, rispettando la volontà del legislatore comunitario ed adempiendo perfettamente ai nostri obblighi di recepimento. Non vedo perché - mi rivolgo anche al ministro Bonino - non prendiamo interamente tutto il dispositivo tutto il dispositivo della direttiva comunitaria e non lo inseriamo direttamente in questo articolo. Noi riteniamo che qualunque ulteriore criterio di recepimento inserito nell'articolo 12

che il decreto legislativo che ne dispone l'attuazione debba contenere clausole o distinguo che rendono più difficile l'immediata sua applicazione. In buona sostanza, signor Presidente, non si vuole un giro

grave problema, perché ci sarebbe una forte possibilità di immigrazione verso l'Italia che andrebbe adeguatamente vagliata; tanto meno in una condizione così possiamo permetterci di non dare indicazioni precise al Governo sul modo di realizzare la direttiva. Vorrei, infine, dire al collega Russo Spena, che ha parlato prima, che per la verità la Costituzione italiana parla di diritti di libertà democratica e l'idea di diritto d'asilo - così come concepito al tempo dei costituenti - si riferisce esclusivamente all'esercizio delle libertà di pensiero, di parola e così via. Stiamo andando molto oltre questo; già la direttiva va oltre questo. L'articolo 12, che stiamo per approvare, va molto oltre questo e quindi credo che proprio da questo punto di vista divenga pleonastico il riferimento all'articolo 10

di ritenere tra i gravi motivi quello della previsione in un diverso ordinamento di un fatto come reato quando tale reato non sia previsto dall'ordinamento italiano e ciò credo che sia molto rischioso. Ci sono Paesi dove l'utilizzo di bevande alcoliche è un reato; allora dobbiamo dare asilo a queste persone. Il nostro Paese potrebbe considerare come reato la non emissione di una fattura fiscale e la stessa cosa vale per gli altri Paesi. Attenzione cioè alla definizione di reato, perché sarebbe una terminologia

di prendere decisioni, per così dire, sull'onda della spinta emozionale, che non necessariamente abbiano un riscontro oggettivo nella necessità dei richiedenti e anche un riscontro oggettivo in ciò che succede in tutto il resto del mondo per casi analoghi.

questo slancio francamente incongruo. Sottolineo che quanto ho sentito mi pare confermi ciò che ho detto precedentemente e cioè che,

solidarietà sociale Paolo Ferrero, del quale apprezzo la sincerità e la schiettezza, che ha parlato anche delle conseguenze in termini di ridisegno della geografia elettorale del Paese grazie ad un afflusso pesante di immigrati con la cittadinanza italiana. Allora anche

Presidente, credo che a questo punto non ci sia la possibilità di concludere il provvedimento. La cosa, purtroppo, è abbastanza grave perché, entrando tra breve nella sessione di bilancio, questo provvedimento slitterà a dicembre, il che non è francamente piacevole. Presidente, mi pare che lei abbia chiesto ai Capigruppo l'orientamento. Se ho capito bene, credo sia il caso di apprezzare le circostanze, visto che ormai sono Presidente, mi sembra di tutta evidenza che tra 20 minuti siamo vicini alle 14 e non c'è nessuna possibilità di votare il provvedimento,

intervenire perché avevo in precedenza già esposto le motivazioni di un mio temporaneo malore che non mi ha consentito di votare. Poiché mi era parso che fossero state tratte da questo elemento puramente numerico valutazioni politiche un po' dispregiative, ho creduto fosse opportuno rimediare a questo. Riconosco che ormai in Aula, per essere credibili, bisogna esibire la cara salma, ma spero che questo non mi succeda. **Mozioni,